di finanza pubblica. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di leggere recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 aprile scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023. Inoltre, il provvedimento, composto di ventitré raccolti in cinque Capi, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica». Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 674 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno della seduta. Passiamo pertanto alla discussione generale relativa alla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale recante

ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

domani approveremo il testo con la maggioranza prescritta anche in seconda deliberazione, il 5 luglio - se non ricordo male - la Camera potrà approvare definitivamente questo importante disegno di legge. Come abbiamo ricordato anche nel corso della discussione che abbiamo tenuto in sede di prima deliberazione,

un elemento importante per garantire la salute psicofisica dei nostri giovani e di tutta la popolazione. L'attività sportiva, infatti, se fatta in modo intelligente, può essere svolta a qualsiasi età. Con questa modifica della Costituzione l'Italia entra nell'elenco ormai abbastanza numeroso dei Paesi dell'Unione europea che hanno inserito la tutela e la promozione dell'attività sportiva o dell'educazione fisica in Costituzione. Ci uniformiamo anche al Trattato di Lisbona che, pur lasciando agli Stati membri questo compito, tuttavia, pone tra gli obiettivi della pone tra gli obiettivi della Costituzione europea, quello di promuovere l'attività sportiva negli Stati membri. Ringrazio tutti i colleghi che hanno votato a favore del provvedimento in prima lettura. Ringrazio il proponente, senatore Iannone, primo firmatario di questo importante disegno di legge che - ricordo - non è giunto al termine nella scorsa legislatura soltanto per l'interruzione anticipata della stessa. E mi auguro che anche in questa seconda lettura il Parlamento, l'Aula del Senato in particolare, nel suo complesso, possa dare un voto favorevole e un apprezzamento positivo al lavoro che è stato fatto, anche grazie al Ministro dello sport che oggi è presente in Aula per seguire il nostro dibattito, e che quindi colgo l'occasione per salutare e ringraziare. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, siamo alla fase finale di un disegno di legge condiviso in modo trasversale da tutte le forze politiche, a testimonianza dell'alto valore dello sport; vi si riconosce la stessa valenza valenza dei diritti fondamentali dell'uomo. Lo sport è considerato alla stregua di un diritto individuale, che porta con sé valori assoluti, come la legalità, la lealtà, il rispetto, il senso di comunità, l'impegno, la condivisione delle regole e il benessere personale. È anche un diritto collettivo, perché un campetto da calcio, Presidente, da basket, da pallavolo o una palestra sono spesso un vero e proprio presidio sociale, ma anche di legalità e di democrazia sul territorio. Non è un caso che ad essere stato modificato sia stato l'articolo 33, a indicarne il valore educativo legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale dello sport. Esprimo soddisfazione perché è stato sancito che lo sport promuove valori direttamente connessi ai principi costituzionali, come l'uguaglianza, l'inclusione e la solidarietà, e che tutto questo è necessario per contrastare ogni tipo di discriminazione, dal razzismo all'omofobia, dal bullismo al cyberbullismo. Esprimo anche un monito, Presidente, affinché tutto questo non rimanga solo un nobile intento, perché il primo approccio che molti dei nostri ragazzi hanno con un campo sportivo avviene nelle palestre delle nostre scuole. Corre l'obbligo allora di porre attenzione al pericolo che molte di queste, soprattutto nel Sud o nelle aree interne, vengano chiuse nel prossimo anno per effetto di calcoli estranei all'onere di questa Repubblica, che deve assicurare l'attività motoria in tutte le sue forme, in modo universale e accessibile a tutti. Infatti, la formula utilizzata, quella di «attività sportive in tutte le sue forme», consente proprio l'accezione più ampia possibile di sport, che sia professionistico, dilettantistico, amatoriale o organizzato; una formula, dunque, che rende merito all'impegno sul territorio di milioni di praticanti, associazioni e volontari, che oggi voglio ringraziare. Tutti abbiamo sottolineato che lo sport è un volano economico che accresce la coesione sociale e la salute collettiva, producendo risparmi per il sistema sanitario; ma servono le risorse economiche per renderlo attuabile e sappiamo che la promozione dello sport è trasversale anche nel PNRR. Anche qui, Presidente, la preoccupazione che opere necessarie non vengano realizzate non è poca. Noi pensiamo che l'inserimento nella Costituzione debba rendere fortemente operativo il Governo nella volontà di attutire i diversi tipi di disuguaglianza nell'accesso allo sport. Diciamo sempre che lo sport deve essere accessibile a tutti. Allora, Presidente, rendiamolo davvero tale.

in un percorso molto veloce, approvare per la seconda volta oggi - come ci auguriamoci e spero all'unanimità - un provvedimento che consentirà allo sport di fare ingresso dalla porta principale nella Costituzione. un'occasione per ribadire alcuni dei concetti e dei principi che a Fratelli d'Italia stanno a cuore, oltre ovviamente a rivolgere un sincero ringraziamento a chi ha portato a compimento questo lavoro che ci deriva dalla passata legislatura e, quindi, al primo firmatario, senatore Iannone, ma anche a tutti i colleghi delle altre forze politiche che hanno saputo fare un passo indietro per trovare un testo unico su uno dei principi fondamentali che tutti quanti riconosciamo. Per aggiungere qualcosa di più al valore dello sport che ci siamo prefissi di inserire in Costituzione,

fatto che manca una reale concezione dello sport come fenomeno sociale e di integrazione con altre politiche di settore che possano essere virtuose per migliorare le altre politiche e non solo sportive. Mi riferisco a quanto può essere considerato e concepito lo sport - non solo in Italia e non solo come valore costituzionale, come ci accingiamo oggi a fare - come principio di riferimento per politiche attive in settori come la sanità

inserendolo anche in progetti scolastici che sono molto importanti fin dalla tenera età. Dispiace ricordare che lo sforzo compiuto dai Governi precedenti di inserire, ad esempio,

certamente tutti vorremmo diventare campioni, ma sappiamo che pochi possono diventarlo. Pensiamo allo sport per stare bene, allo sport per avere un corretto stile di vita e, quindi, ci auguriamo che si arrivi a questo. Colgo anche l'occasione

Ogni palestra chiusa il pomeriggio è un danno per tutta la società, e non solo per quelle società sportive che fanno fatica

parlato molto dell'utilizzo dei fondi pubblici per fare stadi: penso alla polemica del Comune di Firenze, nel quale io sono stato eletto e dove vivo, sull'utilizzo di denari pubblici per lo stadio.

È anche vero che tutti i Comuni, se non le Regioni e lo Stato, aiutano a costruire i nuovi stadi:

anche pubblica, visto che sono fatti con soldi pubblici. Poi certamente ci sarà anche il commercio che dovrà riequilibrare i conti. Non siamo contro il commercio ma, laddove la prevalenza della mano pubblica è sostanziale, vorremmo che ci fosse un ritorno più in termini di socialità e di convivialità,

il disegno di legge Atto Senato 592, di iniziativa governativa, è già stato approvato dalla Camera dei deputati e reca norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022, la cosiddetta riforma Cartabia, ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge, a fronte di questo intervento, che si ritiene di confermare, sono però emersi alcuni problemi, che sono stati evidenziati dalla stampa e dai magistrati competenti, con riferimento a due diversi profili. I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame. Nel merito del provvedimento in esame, l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela, ove ricorrano l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis*.1, comma 1, del codice penale e l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*, comma, 1 del codice penale. In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un comma 6 all'articolo 270-*bis*.1 del codice penale, volto a prevedere che per i reati aggravati dalla circostanza di cui al comma al comma 1, vale a dire dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un comma 5 all'articolo 416-*bis* del codice penale, volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al comma 1 dell'articolo 416-*bis*.1, vale vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio. L'articolo 2 include il delitto di lesioni personali, previsto dall'articolo 582 del codice penale, fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio, qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

nella formulazione vigente, prevede che, in caso di delitto perseguibile a querela di parte, si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il provvedimento modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti non essere prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato, se la querela non è proposta nel termine di quarantott'ore dall'arresto, se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti comunque a effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche in forma semplificata, con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente, che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto facoltativo, in flagranza, possa essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce, nel comma 3, similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, la previsione per la quale, anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale.

volti ad incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza e obbligatorio per le liti procedibili a querela. Le novelle modificano l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 588, sempre del codice di procedura penale, che recano, rispettivamente, la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico. È ben specificare che, nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine delle quarantott'ore per la proposizione della stessa. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Va data menzione, signor Presidente, che gli altri due disegni di legge connessi, l'Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato, e l'Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani, presentano una portata più limitata, intervenendo unicamente in materia di procedibilità di reati, in particolare nei casi di reati aggravati dalla criminalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

onorevoli colleghe e colleghi, come ormai da consolidata tradizione, il disegno di legge governativo prende le mosse da un nostro intervento legislativo. Ormai ci siamo abituati. Purtroppo, però, il vostro è un lavoro di copiatura parziale,

Prima di entrare nello specifico sull'argomento, faccio brevemente una premessa di ordine generale in merito agli emendamenti presentati. Sono stati dichiarati inammissibili emendamenti considerati estranei rispetto all'oggetto del disegno di legge. Lo spirito di una legge - come mi insegnate voi senatori che sedete da generazioni in quest'Aula - lo si considera anche attraverso la lettura, ma soprattutto lo studio dei lavori preparatori. Nella relazione illustrativa del provvedimento si cita a più riprese che l'intento di questa norma è quello di sanare un *vulnus* creato dalla riforma Cartabia. Il relatore, senatore Zanettin, nella dichiarazione di voto in Commissione giustamente, riepilogando le motivazioni sottese al disegno di legge, annuncia che esso è volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia. Io ho riportato testualmente quanto scritto nel Resoconto. Bazoli anche lui interviene in dichiarazione di voto, rilevando che la proposta normativa mira a proporre dei correttivi alla riforma Cartabia. Noi proponiamo emendamenti correttivi alla riforma Cartabia e questi vengono dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Qualcosa non ci quadra. *(Applausi)*. E non erano emendamenti da poco. Con il primo volevamo intervenire al fine di restituire al patteggiamento l'equiparazione alla sentenza di condanna, facendola rientrare nell'applicazione della legge Severino, e con l'altro emendamento sopprimevamo quell'obbrobrio giuridico del concordato in appello. Non mi addentro nel ginepraio della modifica relativa alle condizioni di procedibilità; ne parlerà il senatore Scarpinato, non voglio anticiparvi nulla, ma dico solo: auguri a tutti noi. Parlerò solo di due emendamenti che non abbiamo proprio capito perché nel merito siano stati bocciati. Avevamo previsto l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale e la procedibilità d'ufficio per chi, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, commettesse il delitto di *stalking* o la violazione di domicilio aggravato. Bocciati in Commissione. Perché? Mah. Non eravate quelli a tutela delle donne? Non eravate quelli delle esigenze securitarie? O le esigenze securitarie risiedono solo nel delitto di *rave party*, quando disponevate l'arresto in flagranza dei partecipanti? Ma la cosa - ahimè - più grave non è tanto il comportamento omissivo di non avere approvato emendamenti nostri, bensì quello commissivo, ovvero quanto avete previsto all'interno del testo. L'articolo 3, relativo all'arresto obbligatorio, ribalta infatti totalmente le logiche ed i principi cardine del nostro sistema penale. Non si può anteporre l'arresto ad un atto quale la denuncia, che funge da condizione di procedibilità affinché l'azione penale possa essere iniziata. Si subordina quindi al compimento di un atto futuro ed incerto la libertà personale di un soggetto. In scala di priorità nella salvaguardia dei diritti di una persona, la libertà personale resta uno dei più importanti, se non il più importante. Le esigenze securitarie non possono considerarsi quale diritto tiranno rispetto alla libertà personale, a meno che non si voglia incorrere in una pronuncia di incostituzionalità. Quindi resteremo vigili anche su questo punto. I punti appena evidenziati relativi al disegno di legge in esame attengono a questioni sulle quali il legislatore ha ancora il potere di intervenire. Io, da buona napoletana, sono e sarò sempre ottimista, quindi siamo fiduciosi sul anche perché questo non è un decreto-legge, ma un disegno di legge di iniziativa governativa, quindi non deve essere approvato in sessanta giorni e ci può essere un supplemento di riflessione. Fermatevi, valutate e poi nel merito, in caso, bocciate; non bocciate per poi pentirvi di non aver valutato. *(Applausi)*.

a procedibilità d'ufficio sono quelli ritenuti più gravi, per cui, appresa la notizia da parte dell'autorità giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga una querela. I reati a querela di parte sono invece quelli ritenuti meno gravi, per cui è necessaria una querela della persona offesa. La querela contiene la specifica richiesta della persona offesa di ottenere la punizione del soggetto che ha commesso il fatto illecito penalmente rilevante nei suoi confronti. Quindi è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato o il suo legale rappresentante esprimono la volontà che si proceda per punire il colpevole. È prevista dall'articolo 336 del codice di procedura penale e riguarda ovviamente i reati che non sono procedibili d'ufficio. Fino ad oggi, quindi, procedibilità d'ufficio e procedibilità a querela erano le due categorie utili a soppesare l'importanza delle violazioni di legge penale. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale che sono stati invece perseguiti dalla riforma Cartabia, abbiamo assistito nel corso della scorsa legislatura alla decisione parlamentarizzata di un ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nel libro secondo e terzo del codice penale. Quindi con la riforma Cartabia si amplia la portata dei casi nei quali si condiziona la repressione penale di un fatto astrattamente offensivo alla valutazione in concreto e alla sovranità della persona offesa. Tale opzione, a dire il vero, era già stata inaugurata per la prima volta con una più poderosa e ampia normazione, che era la legge n. 689 del 1981, proseguita con la legge n. 205 del 1999. Questa scia normativa è tipica di una tendenza alla privatizzazione, detta anche patrimonializzazione della tutela penale, che denota l'importanza crescente della funzione cosiddetta selettiva della querela-selezione; ovverosia la querela diventa lo strumento con il quale, ampliando o diminuendo la forbice di operatività di questa facoltà, si rende più o meno incidente il ricorrere di contestazioni che poi sfociano in un procedimento. In altri termini, la querela diventa lo strumento politico-criminale volto a contemperare la superfluità della pena in concreto. Questa linea di pensiero è stata quella con la quale la riforma dell'ex ministro Cartabia ha in qualche modo rimesso in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale, ritenendo che vi fossero un'ipertrofia della legislazione penale e un numero sempre più insostenibile di procedimenti a cui porre rimedio. Si disse che si doveva valorizzare la procedibilità a querela e che si sarebbe in quel modo ridotta in modo corrispondente l'area della procedibilità d'ufficio, con una strategia finalizzata a migliorare l'efficienza del processo penale al fine di centrare gli obiettivi del PNRR, con una riduzione stimata del 25 per cento dei tempi medi del processo penale. Ovviamente, quando si pongono in essere queste operazioni di taglio orizzontale, ci si accorge con il tempo che, per alcuni tipi di reati,

come la minaccia o la lesione, possono essere collocati all'interno di una più articolata operatività di soggetti criminali che lavorano all'interno di strutture che hanno una una propria regolamentazione, che da un punto di vista giudiziario può essere facilmente riconoscibile. È per questo che, con il testo in esame in esame oggi pomeriggio, andiamo a correggere quelle storture che abbiamo ritenuto critiche della riforma Cartabia. Lo facciamo all'articolo 1 - lo ricordava il relatore ponendo mano agli articoli 270-*bis*.1 e 416-*bis*.1 del codice penale, che riguardano rispettivamente le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e le associazioni di tipo mafioso, che fanno appunto dell'intimidazione e dello strumento della violenza un vincolo di assoggettamento e di omertà, con il quale possono, attraverso una miriade di

di "arrestare" (in termine atecnico e in termine tecnico) il soggetto criminale che magari avesse agito nell'ottica di una strategia di ordine criminale. Ma non solo: qualora la persona offesa fosse presente al momento al momento dell'arresto, garantiamo il diritto di procedere oralmente con la sua manifestazione di volontà.

possibilità, che lo Stato vede come strumento certamente social-preventivo, per tutta una serie di condotte che riteniamo assolutamente preoccupanti

pienamente soddisfatti di questa proposta che, nel testo che abbiamo adottato, porta la firma del ministro della giustizia Nordio, che ringraziamo per questo atto di sensibilità che mette nuovamente il nostro Paese nelle condizioni di porre un freno a determinate condotte riprovevoli e assolutamente estranee alla nostra cultura e al nostro modo di vedere la giustizia nel nostro Paese. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando.

Avevamo iniziato questa discussione con grande clamore sui *media*, anche suscitato da esponenti politici, con un attacco ad alzo zero alla riforma Cartabia, addebitandole guasti incredibili che, per fortuna, non solo non si son verificati, ma non si potevano verificare, perché era evidente che anche persone in custodia cautelare per reati legati alla mafia non sarebbero certamente uscite a causa della procedibilità a querela. Vediamo con un certo sollievo che anche quello del Governo è un intervento assolutamente chirurgico e comunque conferma la validità di alcune scelte di fondo della riforma. Peraltro, l'intervento raccoglie proposte di diverse forze politiche, tra cui anche la nostra. D'altra parte,

dell'intervento penale. Ecco, mi corre l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni su questo. Innanzi tutto, le questioni su cui interviene questo disegno di legge in modo chirurgico esistevano già precedentemente alla riforma Cartabia ma, ovviamente, ampliando il sistema dei reati perseguibili a querela, sono venute più all'attenzione.

da prima non erano procedibili d'ufficio reati che erano perseguibili a querela. Lo stesso dicasi per il tema dell'arresto in flagranza. Il punto qual è?

di difendere il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è un principio cardine nel nostro ordinamento, al quale è legato ovviamente anche quello dell'autonomia e dell'indipendenza, perché non esiste un potere discrezionale che non sia vincolato da un altro potere, vuoi elettivo, vuoi di sottoposizione all'Esecutivo. Si fa una scelta precisa, facendosi carico del tema dei temi, cioè di un eccessivo carico di domanda penale a risposta di qualsiasi problema sociale. Da questo punto di vista, l'esordio

querela; una scelta di sistema, accompagnata da una grande attenzione alla giustizia riparativa, laddove la persona offesa non viene abbandonata,

un luogo in cui viene sanata l'offesa, la possibilità di trovare questa riparazione come alternativa ai tre gradi di giudizio nel processo penale. È una scelta di sistema molto chiara che vuole farsi carico dei problemi e che non vuole lasciare soli i cittadini. La scelta della perseguibilità a querela, accanto a un grande intervento di giustizia riparativa e a una serie di elementi introdotti in tutto

Perché, quando c'è l'aggravante del metodo mafioso e l'aggravante di terrorismo, il reato non è più perseguibile a querela? Perché c'è un interesse anche prevalentemente di natura pubblica; non è un fatto che appartiene solo al privato; c'è ovviamente la questione dell'intimidazione, ma il fatto è che ha anche una diversa collocazione nella scala dei valori. Vi è un punto più delicato su cui avevamo proposto anche noi degli emendamenti: ad esempio, quando sussiste la dissociazione dai reati, secondo noi doveva comunque permanere la procedibilità d'ufficio. Questo suggerimento non è stato raccolto, a proposito di tutela della sicurezza e dell'essere molto attenti quando c'è un certo tipo di offensività.

libertà personale, prima ancora che sia stata presentata una querela, e la sicurezza dei cittadini. È stato trovato un punto di equilibrio:

vale per l'intervento sulle lesioni, quando è stata emessa una misura di prevenzione. In sostanza, si poteva sicuramente

eminentemente economicistiche, ma su una scelta di sistema per una maggiore tutela dei cittadini, non per una privatizzazione della tutela, laddove si intende che l'intervento dello Stato non è

una procedura di accompagnamento e di presa in carico della persona offesa non necessariamente attraverso tutto l'*iter* processuale. Naturalmente noi avremmo voluto molta più giustizia riparativa di quella che c'è nella riforma, ma sappiamo anche che tale riforma è il frutto di un preziosissimo lavoro che ha visto l'approvazione della quasi totalità delle forze presenti in Parlamento. Su questioni così rilevanti, rilevanti, noi lo riteniamo un risultato importante, non una mediazione al ribasso. Ora, ci preme sottolineare che questa che questa riforma ha una portata molto grande, che implica un intervento importante nella visione che mettiamo in quella che un po' riduttivamente definiamo l'organizzazione della giustizia.

non vediamo ancora nessun segnale, anzi vediamo dei segnali in senso opposto: moltiplicazione di reati, proclami di continui interventi di riforma di cui non si intravede neanche una bozza

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti sappiamo, la riforma Cartabia, entrata in vigore il 22 dicembre 2022, aveva l'obiettivo di accelerare la durata del processo e ciò anche attraverso la deflazione e la digitalizzazione del procedimento. Proprio questa mattina la Commissione giustizia era alla procura di Roma e ci siamo soffermati su questo aspetto, ricevendo degli spunti interessanti sui quali lavorare. Tornando sull'accelerazione, questa finalità emerge chiaramente anche dall'intervento sull'impugnazione che viene dichiarata improcedibile qualora il giudizio di appello o di cassazione si protraggano eccessivamente. Sotto il profilo della deflazione, la riforma ha operato sulla procedibilità per alcuni reati contro la persona e il patrimonio, stabilendo che siano perseguibili soltanto a querela di parte, querela necessaria anche per l'arresto in flagranza e il mantenimento delle misure cautelari. Perseguibilità a querela significa che senza l'iniziativa di parte il procedimento non viene mai ad esistenza, ma il legislatore è come l'ingegnere che progetta un motore: talvolta il meccanismo che appare ben congegnato, una volta messo in azione può mostrare difetti, soprattutto quando lavora in condizioni critiche e rende quindi necessarie messe a punto e talvolta modifiche per eliminare i vizi di funzionamento. Così la riforma Cartabia, una volta applicata, ha rivelato difetti operativi che hanno richiesto correzioni immediate. È emerso, infatti, da un lato che la persona offesa non è sempre in grado di scegliere liberamente se sporgere querela oppure no e dall'altro che non sempre la persona offesa può essere reperita immediatamente. Sotto un altro aspetto, si è verificato che a chi aveva commesso un reato di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, in seguito all'introduzione della perseguibilità a querela, sono state revocate le misure cautelari. L'intervento è stato immediato. Il 19 gennaio, quindi dopo meno di trenta giorni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, il Governo ha corretto il meccanismo attraverso il disegno di legge che oggi è in esame in quest'Aula. Questo disegno di legge stabilisce che nell'ipotesi in cui il reato sia aggravato da mafia o terrorismo si proceda d'ufficio e si possa procedere ad arresto in flagranza anche in mancanza di querela. Un intervento correttivo quanto mai importante, ad esempio, quando si verificano i furti di cui all'articolo 380, comma primo, lettera *e)* del codice di procedura penale, commessi in orario notturno e la vittima non sia rintracciabile, oppure quando vi sia la necessità di perseguire alcuni reati, quando siano commessi in ambito mafioso, in cui la vittima spesso non sporge querela per paura di esporsi a vendette e ritorsioni. Risposta immediata a un problema urgente: questo è il metodo che il Governo ha seguito, affinché il *summum ius* non si tramuti mai in *summa iniuria*. Dichiaro chiusa la discussione generale. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

questo tema questa settimana anche con tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione proprio a Ravenna, insieme al presidente della Regione Bonaccini e addirittura il ministro Musumeci è venuto a parlare a Faenza per cercare di capire come intervenire. Ovviamente in questo